una sospensione dei controlli proprio sulla sicurezza e sulla salute sul luogo di lavoro. Tale sospensione è stata introdotta con il maxiemendamento che ha finito per costituire il testo dell'articolo unico della legge finanziaria.

per confermare o meno all'Aula del Senato se al vice ministro Visco fossero state riconsegnate - so di usare un termine improprio,

Presidente, chiedo come sia possibile accantonare l'articolo 7, che parla delle tariffe, e passare all'articolo 8, che parla della copertura finanziaria.

all'inizio dell'esame degli emendamenti, una domanda che mi sembrava avesse bisogno di una risposta.

su indicazione della Commissione, sono state inserite alcune parole, alla fine dell'emendamento 9.0.1 (testo 2) che danno un completamento e una maggior comprensione dell'articolo. Bene.

«Sostituire l'articolo con il seguente: Articolo 8 (Oneri finanziari): 1. «I nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto sono posti a carico del bilancio della regione Campania».

riformulare il testo di un emendamento non solo con delle aggiunte e con delle correzioni che lo rendano più comprensibile? Avendo

le preciso che, in via generale, è nella piena disponibilità di ciascun presentatore la potestà di riformulare le proposte emendative a propria firma. In particolare, le modifiche apportate al testo della proposta emendativa in questione attengono alla copertura finanziaria e conseguono direttamente dal parere espresso dalla Commissione bilancio sull'iniziale formulazione dell'emendamento medesimo. Per queste ragioni, alla luce di una prassi costante e mai posta in discussione, la riformulazione dell'emendamento in questione è da considerarsi pacificamente ammissibile. Quindi, possiamo andare avanti, senatore.

il sottoscritto può, anche in Aula, cambiare il testo di un emendamento, riformulandolo, anche stravolgendolo completamente, come è stato fatto in questo caso.

Non abbiamo fatto, come lei ha visto, pratica ostruzionistica in questa occasione; anzi, sia in Commissione sia in Aula, abbiamo mostrato di voler costruire un testo il più compatibile possibile con il nostro ordinamento.

Signor Presidente, se lei ha intenzione di sospendere la seduta, allora le vorrei chiedere di trasmettere immediatamente alla Commissione bilancio il testo di un emendamento riformulato che noi non abbiamo ancora esaminato, ma che certamente dobbiamo riesaminare. Se lei sospende per venti minuti e mi autorizza a convocare la Commissione bilancio,

di innovazioni che hanno rilievo finanziario sta diventando veramente molto difficile. Se quindi c'è un ulteriore emendamento, ce lo diano, se non c'è, non ce lo diano e finiamola lì.

cioè lo scioglimento del Comune. Se però viene nominato un commissario che adotta come tale la delibera che avrebbe dovuto adottare il Consiglio comunale, non c'è più ragione di sciogliere lo stesso, perché la delibera c'è e c'è la norma che stabilisce la tariffa, come prevede la prima parte dell'articolo 7; quindi, non vedo perché venga richiamato l'articolo 141, comma 1, che è dedicato allo scioglimento del Consiglio comunale. Leggendo la norma, sembrerebbe

non c'è alcuna anomalia perché si replica una procedura utilizzata e diffusa in casi simili, non ultima l'evenienza che il Consiglio comunale non adotti nei termini previsti il bilancio, nel qual caso si nomina un commissario *ad acta* che adotta il bilancio, ma si avvia la procedura di scioglimento per grave violazione di legge. È evidente che con la proposta del Governo intendiamo assimilare la mancata previsione della tariffa corrispondente ai costi del Comune ad una grave violazione di legge; altrimenti, se non c'è una sanzione severa, diciamo la verità, manteniamo la situazione esistente da questo punto di vista, e non voglio dire altro. La risposta mi pare chiara, a parte il giudizio di merito. Un minuto, senatore Pastore, sono finiti i tempi. per una delibera che comunque viene posta in essere dal commissario *ad acta*. Quindi, si aggiunge questa sanzione che è del tutto eccezionale. Io non sono d'accordo, ma mi fa piacere che sia chiaro in quest'Aula a quali conseguenze può portare

Mi perdoni, Presidente, l'articolo 7 non riguarda solamente la questione esposta dal senatore Pastore, ma anche una delle problematiche fondamentali ai fini della copertura

che, attraverso l'articolo 7, si voglia scaricare sui cittadini della Campania tutto il costo dell'operazione emergenza. Infatti, come diremo anche nel corso dell'esame dell'articolo 8, signor Presidente, il Governo si è ostinato a non volerci rappresentare l'entità di questo costo; ci ha solamente indicato quali erano le disponibilità nei capitoli di bilancio della Protezione civile; ci dice poi che c'è una clausola di invarianza della spesa, ma non quanto costa l'operazione e ogni volta che si aggiunge un costo

alla clausola di invarianza della spesa. Ciò significa che quella spesa aggiuntiva dovrà uscire dalle previsioni dell'articolo 7, cioè dalle tariffe che i Comuni dovranno adottare

spese. La vera emergenza, signor Presidente e colleghi, non sono i rifiuti in Campania, ma l'atteggiamento di questa maggioranza e di questo Governo che non vogliono disporre le somme necessarie per ovviare all'emergenza. *(Applausi dal Gruppo* *FI).* Questa è la vera emergenza e la vogliono caricare sulle spalle dei cittadini campani;

la ringrazio della possibilità di parlare. Intervengo solo per dire che ringrazio il collega D'Andrea che ha spiegato, in modo ineccepibile e corretto, che è chiaro - e i colleghi del centro-sinistra lo devono avere chiaro che, in mancanza della delibera di aumentare le tariffe, si scioglie il Consiglio comunale. Avevate creduto di aggirare questo problema ed esso rimane. È bene che si sappia che si sciolgono tutti i Consigli comunali della Campania che non adottano queste delibere. È una cosa mostruosa, ma è bene che lo sappiate. Il Governo ha risposto in modo preciso;

il collega Pastore ha espresso il dubbio che con la nuova formulazione non si sciolgano i Consigli comunali e al contrario il senatore D'Onofrio è preoccupato che li si sciolga. La verità è che le tariffe non saranno pagate dai cittadini. Per ciò che riguarda l'emergenza, questo è stato precisato all'articolo 8 del disegno di legge; è chiaro che con i fondi a disposizione del commissario si coprirà l'emergenza fino al 31 dicembre; ciò che verrà dopo, che è l'ordinario (ed è un ordinario dovuto anche alle positive modifiche introdotte dalla Commissione), sarà fatto dai Comuni, come è giusto, che lo pagheranno escludendo i costi dell'emergenza dalle loro tariffe. Ciò, peraltro, serve finalmente a fare in modo che i Comuni facciano la raccolta differenziata, che rappresenta un grande valore economico.

all'anticipazione per i Comuni della Campania del meccanismo tariffario previsto tra due anni sul piano nazionale. E ci troviamo di fronte, in alcuni Comuni della Campania, al passaggio dal meccanismo della TARSU al meccanismo della TIA, cioè dalla tassa alla tariffa, e cioè dalla possibilità di copertura della tassa per l'85 per cento all'obbligo di copertura della tariffa del 100 per cento. Deve essere chiaro che c'è, di per sé, una straordinaria impennata tariffaria per i cittadini della Campania: al di là dell'emergenza o dell'ordinario, di fatto c'è un meccanismo di questo tipo. Allora, vorrei dire al senatore Castelli, che giustamente fa determinate considerazioni (e lo capisco), che sarebbe giusto dire con chiarezza che questo provvedimento deve avere una copertura federalista; la Campania si deve assumere le responsabilità del suo fallimento *(Applausi deve determinare l'utilizzo finalizzato ad affrontare questa emergenza, anziché a consolidare il potere clientelare e lottizzatorio del centro-sinistra! *(Applausi dai

si continua a dire che i costi, al di là di quanto sostiene il senatore Tecce, li pagano i cittadini campani. Mi piacerebbe sapere dal sindaco Mastella e dal senatore Pecoraro Scanio se intendono far pagare ai cittadini campani il disastro e il dissesto esistenti. Lo andranno a spiegare loro ai propri cittadini.

è possibile individuare una sorta di clausola di salvaguardia per il cittadino? Capisco la riflessione della 5a Commissione e del presidente Morando a proposito della copertura,

per quale motivo, visto che c'è un meccanismo tariffario, devo pagare per un servizio che non ricevo? Aggiungo che sta accadendo questo, giudici di pace, che certo non sono la Cassazione, hanno già affrontato in via di contenzioso questo tema ed hanno riconosciuto ai cittadini non solo la possibilità di pagare il 40 per cento, ma anche il risarcimento del danno.

per stabilire un principio che dica che, se non c'è il servizio, il cittadino non deve pagare.

momento che da molti colleghi, anche dell'opposizione, è stato sollevato il problema della copertura degli oneri derivanti dall'approvazione del provvedimento in esame. Questa è stata anche la mia preoccupazione nella stesura del testo originario dell'emendamento in modo da rafforzare la clausola di invarianza della spesa a carico del bilancio dello Stato.

nel senso di prevedere il monitoraggio continuo degli oneri e la presentazione di una relazione bimestrale al Parlamento in merito all'utilizzo delle risorse già disponibili sulla contabilità speciale del commissario. onorevoli colleghi, non è stanziare ulteriori risorse ma controllare come vengono spese quelle già previste. Ricordo la relazione della Corte dei conti in ordine all'entità 850 milioni di euro di risorse destinate alla sola Campania e all'utilizzo delle risorse assegnate alle gestioni commissariali negli ultimi dieci anni. La Corte è stata impietosa nel denunciare sprechi ed omissioni di vigilanza. Credo che un controllo continuativo sia doveroso per rendere conto ai cittadini, non solo campani ma italiani tutti, come vengono spese le risorse della fiscalità generale.

Presidente, le ribadisco il mio disappunto per il fatto che in quest'Aula sia stato accolto questo emendamento quando i termini di presentazione erano già scaduti. già scaduti. Mi meraviglio di come il collega Morando, presidente della 5a Commissione, non abbia dichiarato l'originario emendamento 8.100 improponibile, perché va assolutamente contro lo spirito di questo vostro decreto. Un suggerimento soltanto vorrei permettermi di dare: invece di fissare una rivisitazione completamente opposta, come è stato fatto in quest'occasione, suggerirei al relatore

Presidente, abbiamo presentato questo emendamento perché permane l'assoluto silenzio del Governo in ordine alla stima delle spese relative agli interventi previsti da questo decreto. Il Governo, con la clausola d'invarianza della spesa, ci rinvia alle disponibilità esistenti in quei capitoli e non ci dice a quanto ammonteranno quelle spese e quindi non sappiamo se quei capitoli saranno capienti o meno; riteniamo che quei capitoli non siano capienti capienti e che quindi ad un certo punto l'attività del commissario per l'emergenza dovrà essere sospesa perché avrà esaurito fondi palesemente non capienti, tant'è che la Commissione bilancio non lesina pareri contrari ogni qual volta si propone un ulteriore adempimento a carico del commissario per l'emergenza. Allora, la cosa più onesta che il Parlamento ed il Governo possono fare è di stanziare una cifra vera per questa emergenza, commisurata alle effettive necessità. È per questo che noi chiediamo che ciò avvenga tramite questo emendamento. Se non passa questo emendamento l'attività del commissario si blocca nel giro di poche settimane o, come abbiamo purtroppo paventato e dimostrato dianzi, il costo lo pagheranno i cittadini della Campania.

Presidente, le avevo chiesto la parola sull'emendamento precedente. Voglio soltanto lasciare questo messaggio telegrafico: a mio avviso, a mio avviso, l'emendamento che abbiamo votato in precedenza rinvia alla contabilità speciale,

capisco, ma non sono d'accordo - noi stiamo travolgendo un'innovazione regolamentare che adottammo nella scorsa legislatura, a mio avviso, di grande pregio che non andrebbe abbandonata. Il parere contrario della 5a Commissione ai

per trasformarlo semmai in ordine del giorno perché il senso è condivisibile, ma è un obiettivo che va ovviamente istruito operativamente. Nel caso non fosse trasformato in ordine del giorno, il parere è contrario.

In sostituzione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, il Commissario delegato adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

In sostituzione del piano regionale si commissaria la Regione, poi si scrive però che si deve sentire il commissario per la bonifica. si commissaria Bassolino come presidente della Regione e si sente come commissario per la bonifica; ma veramente questo articolo non può essere votato da nessuno. *(Applausi dai

Presidente, abbiamo presentato un emendamento per far coincidere la figura del Commissario delegato con quella del Commissario per la bonifica. Il senatore Matteoli ha testé svolto correttamente il riferimento all'impostazione dell'articolo 9: se si commissaria il Presidente della Regione e lo stesso Consiglio regionale in relazione al piano regionale, non si capisce per quale motivo debba esservi il concerto del Commissario per la bonifica. Mi pare che nella logica dell'impostazione del provvedimento, l'emendamento 9.20/4, che elimina quel passaggio e quel concerto, dovrebbe essere votato proprio nell'impostazione consequenziale dell'articolo.

presente che solo nelle commedie dell'arte era lecito aspettarsi che si potesse commissariare addirittura una realtà istituzionale com'è la Regione, con il suo Consiglio regionale e la sua Giunta, poi far risorgere da queste ceneri un personaggio come Bassolino, una specie di entità disincarnata rispetto alla realtà regionale, ridandogli quei poteri che vengono avulsi alla Regione. *(Applausi dai Gruppi FI e AN)*. Credo, signor Presidente, che sia un fatto profondamente incostituzionale, perché viola la realtà che lega la Regione ai suoi doveri, alle sue funzioni e alla sua rappresentanza, attribuendo a un commissario il potere che le viene così sottratto. Non so, cari amici, se possiamo sopportare, nel nome di un'emergenza, l'emergenza vera, che è quella di distruggere la rappresentanza popolare per affidarla a un commissario, chiunque egli sia, Bassolino compreso.

Ne ha facoltà. D'ALI' *(FI)*. Signor Presidente, ancora una volta ci troviamo di fronte ad una variante proposta all'ultimo momento dal relatore che comporta maggiori spese.

oneri, incombenze e prescrizioni per il Commissario, più presto i soldi finiranno, più presto si ricorrerà alla tassazione straordinaria e, in maggiore misura, per i cittadini della Campania. Questo vezzo, ripeto, deriva dal fatto che ancora nessuno ha voluto chiarire l'entità esatta dei costi dell'emergenza e delle operazioni previste da questo decreto, rifugiandosi dietro l'esistenza di un fondo della Protezione civile, che dovrebbe essere interamente utilizzato e che è quantificato in 12,3 milioni di euro, che sono palesemente insufficienti per ottemperare a tali prescrizioni. Vorrei sapere dal Governo cosa ne pensa il Commissario delegato di questa ulteriore prescrizione che gli impone prescrizione che gli impone di attrezzare, entro 90 giorni, almeno un sito con le caratteristiche qui individuate, sapendo che quest'operazione è di impossibile fattura e di enorme costo. Ancora una volta ci nascondiamo dietro il dito dell'invarianza di spesa; ancora una volta poniamo una condizione perché l'emergenza rimanga tale, perché gli interventi non possano essere assolti, perché i cittadini campani debbano pagarne lo scotto.

l'intervento del presidente Sodano

Se il presidente Sodano è d'accordo sull'impostazione iniziale, potremmo votare l'emendamento fino a «smaltimento dei rifiuti». Praticamente, il testo reciterebbe: «Le Province provvedono entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore

si disturbasse ad esprimere un parere in proposito, perché ritengo che sia giusto che lo faccia.

al senatore Matteoli che il problema sta nel principio che, approvando questo emendamento, andrebbe contro tutto quello che abbiamo detto, anche voi, durante la discussione sia in Commissione che qui. Stiamo votando con qualche difficoltà, ma con la responsabilità di chi deve affrontare una questione veramente drammatica, un decreto che prevede una serie di emergenze, ma nessuno di noi pensa che la gestione dei rifiuti si possa risolvere solo collocando impianti.

ed è finalizzato a contrastare il fenomeno del traffico illecito. Credo che potrebbe benissimo essere accolto in quanto determinerebbe una maggiore serenità

Gruppi sono esauriti, ma dato il rilievo dell'argomento che abbiamo affrontato e anche, malgrado le polemiche che vi sono state nel dibattito,

comprendo anche il disagio, non solo dei colleghi di maggioranza che con me sostengono questo decreto-legge alla cui conversione annuncio voto favorevole, degli stessi colleghi dell'opposizione che, per l'ennesima volta, vedono portare in Aula un tema che riguarda l'emergenza rifiuti in Campania.

che non è altro che seguire con determinazione e intelligenza le indicazioni della Comunità Europea. Si tratta quindi di fare esattamente il contrario di come si è proceduto fino adesso in Campania, anche con chiare responsabilità delle istituzioni che hanno governato, e che ha portato a considerare la discarica come unico strumento di gestione dei rifiuti.

proprio perché le istituzioni vivono ancora un momento che definisco benevolmente di convalescenza, deve consistere in uno strumento chiaro, spiegabile ai cittadini, ordinario, già esistente nelle norme e nelle leggi italiane, che peraltro collabora ad eliminare uno dei tanti enti intermedi di intermediazione e di distorsione della gestione delle risorse che in Campania si sono moltiplicati e di cui il commissariato è la massima espressione.

e Province si mettano assieme per lavorare lungo tre direttrici: piano integrato dei rifiuti, che veda alti livelli di raccolta differenziata, impianti di trattamento e impianti finali di smaltimento a norma con le migliori tecnologie possibili; piano di bonifiche correlato al piano integrato dei rifiuti; rifiuti; possibilità di sfruttare i fondi europei, di cui la Regione Campania disporrà in maniera copiosa dal 2007 al 2013, per dare il senso a quelle comunità che avranno l'onere di avere insediamenti di impianti e di tecnologie di avere anche delle opportunità di sviluppo. L'unico modo per andare avanti ed evitare proteste, a volte legittime, a volte guidate solo della piazza e non dalla conoscenza dei fatti e sulla base di una informazione corretta, è che tutta la comunità campana abbia il senso insieme di fare uno sforzo per

siamo ad un punto cruciale per far fronte alla situazione drammatica dello smaltimento dei rifiuti della Campania e, dunque, non possiamo - proprio noi - determinare uno stallo del contesto emergenziale. A noi il compito di dare una stangata all'emergenza, supportando l'azione di Bertolaso che, ancora una volta, va agevolata e spianata in ogni modo, affinché la nostra *Terra Felix* esca definitivamente da questa *impasse*. Forse è ancora caro il prezzo da corrispondere a fronte della normalità gestionale, giacché si tratta di riaprire alcune discariche già al tracollo - Acerra -piuttosto che realizzare nuovi luoghi di sversamento - Terzigno - nel cuore del Parco nazionale del Vesuvio. Comunque, se servirà a vedere la Campania riemergere da quest'onta, che la vede da più di 14 anni succube delle ecomafie e dell'irresponsabilità, se le soluzioni alternative saranno rapide allora possiamo - ancora una volta - soprassedere sui mezzi, perché il fine è assicurato. Ora è tempo in cui le forze devono essere convogliate a conseguire un risultato positivo. È il caso di sottolineare - per chiarezza e correttezza - che questo modo di procedere è costato tanto ai cittadini di terre già vessate. Mi è d'uopo una breve precisazione che serve a comprendere come proprio io da parlamentare incoraggi la conversione del decreto odierno, nonostante abbia visto svanire il tentativo di evitare danni maggiori alle cittadinanze interessate, sia sotto il profilo sanitario

che contiene il serio impegno del Governo a valutare l'inopportunità dell'eventuale ulteriore utilizzo del sito provvisorio di stoccaggio localizzato

dell'Esecutivo rappresenta un segno tangibile per il futuro dei cittadini di Acerra, nell'attesa che questi, così come tutti gli altri cittadini campani, non debbano più pagare le tragiche conseguenze delle gestioni emergenziali e che si passi una volta per tutte alla gestione ordinaria dei rifiuti nella Regione. Dunque, se il presente decreto-legge non è finalizzato solo momentaneamente a fronteggiare una situazione difficile che poi resta tale - e si spinge a mettere in atto nella Regione un appianamento definitivo dello smaltimento dei rifiuti, allora si può stringere i denti e proseguire il sentiero di scelte impopolari, quanto meno risolutive. Se si tratta di apportare un intervento coerente, che garantirà il passaggio alla gestione ordinaria dell'«inferno ambientale campano», allora siamo tutti d'accordo. Se così non fosse, viceversa, mi domanderei come sia possibile che il Governo dichiari, ad esempio, lo stato di emergenza socio-economica in relazione all'inquinamento ambientale da diossina accertato nel territorio del Comune di Acerra e, contemporaneamente, il commissario straordinario Bertolaso, continui a localizzare siti di stoccaggio nel medesimo territorio che riguardano milioni di tonnellate di rifiuti non differenziati e non trattati. Allora dovrei constatare che siamo ad un dichiarato fallimento, che non ammette via d'uscita, immersi in un mare di incapacità ed irresponsabilità. Per fortuna è ipotesi lontana dal mio - spero nostro - ottimismo. Ottimismo che nasce dalle novità del provvedimento, che intensificherà i controlli sulla raccolta differenziata, grazie all'azione dei subcommissari e delle commissioni di recente nomina e impegnerà attivamente i Presidenti di Provincia, cui sarà affidato un ruolo istituzionale concreto, con l'obiettivo di stabilire un filo diretto con il territorio per scelte di rapida soluzione, individuare siti di sversamento in collaborazione con cittadini ed associazioni interessate. In poche parole, l'ottimismo che mi porta a dichiarare il favore dell'Udeur

che il Governo ha emanato sotto la spinta della necessità e dell'urgenza. Mi sembra quasi di vivere un *déjà vu* o forse posso dire che sia un ricordo lungo ben 14 anni e che ci ha riuniti anche di recente.

La situazione oramai può facilmente definirsi di cronica incapacità a far funzionare un sistema di smaltimento come accade in tutto il resto d'Italia, salvo qualche prestigiosa realtà. Una situazione di cronica inefficacia a cui si cerca di porre rimedio con provvedimenti tampone, mascherati dall'emergenza. Non potete chiederci, a questo punto, di condividere un ulteriore provvedimento con i connotati della necessità e dell'urgenza. Alla base di questo ennesimo decreto rifiuti vi è una lunghissima serie di errori madornali e di cattive, successive, strategie messe in campo. La gravità del problema dei rifiuti si aggiunge come un macigno alle mille problematiche di una Regione già martoriata, purtroppo, a causa di un malgoverno di ormai lunga durata della Sinistra, sia a livello regionale, sia a livello comunale, nel capoluogo campano, la quale si è resa colpevole, con gesti avventati e provvedimenti successivi poco incisivi, di un vero e proprio disastro ambientale. Tra l'altro, volevo domandare ai colleghi DS se al loro interno ogni tanto chiedono conto a questi due autorevoli loro rappresentanti (DS e Margherita), una sindaco di Napoli e l'altro Presidente della Campania, perché oggettivamente i cittadini tra breve assalteranno le due sedi della Regione e del e del Comune di Napoli, dal momento che è insopportabile quella situazione; tanta clientela e poche soluzioni, forse anche quelle figlie di un sistema elettorale, come quello per l'elezione del Presidente della Regione e del Sindaco, sbagliato. «Abbiamo un nuovo viceré», lo hanno titolato tutti i giornali, ma voi parlamentari sotto questo punto di vista sembrate impermeabili. Non fa Non fa eccezione la vicenda di cui stiamo parlando oggi, anzi è il fiore all'occhiello della Sinistra campana. Accanto al problema già grave dei rifiuti, il suolo campano si trova a dover quotidianamente combattere contro altre gravissime piaghe come quelle della criminalità organizzata, che miete vittime anche tra la popolazione della città, e del *deficit* pubblico; problematiche concatenate tra loro in un vorticoso sistema che si autoalimenta grazie anche all'inerzia e alla compiacenza dell'*establishment* politico della Regione. Anche per questa volta il Governo corre ai ripari proponendo a noi e ai cittadini italiani provvedimenti di urgenza, senza mai arrivare, tuttavia, a mettere in discussione l'operato degli amministratori locali di Sinistra, che avrebbero dovuto provvedere quotidianamente alla corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti. Siamo di fronte all'ennesima situazione a cui questo Governo, in poco più di un anno, ci ha ormai abituato: emergenza al posto di serie riforme strutturali volte alla eliminazione delle cause, cioè lotta alla camorra e un meditato piano impiantistico per lo smaltimento dei rifiuti accumulati. Come non criticare poi la scelta di individuare siti da destinare a luogo di discarica all'interno di un Parco nazionale come quello vesuviano, che porterà giustamente e inevitabilmente la Comunità europea ad aprire un procedimento di infrazione. Si tratta di un provvedimento che non riesce a dare ossigeno ad una Regione che muore soffocata tra i fumi dei rifiuti, come soffocata è la sua economia la sua immagine, anche a livello internazionale. Il resto dell'Italia è così costretto ancora oggi ad assistere a tale catastrofe non potendo disporre che solo del proprio sdegno. Allora mi chiedo, e mi rivolgo anche ai colleghi della maggioranza: possiamo noi oggi qui rimanere ancora in silenzio, assecondando e così tacitamente avallando coloro che del silenzio e del malcostume della corruzione hanno fatto uno stile di governo del territorio? Ecco perché ci opponiamo, ancora una volta e con sempre più forza, a questi continui, inutili e deleteri provvedimenti tampone.

quando si ha una malattia molto grave, quasi terminale,

addirittura a rimedi magici, a pozioni, oppure, quando va bene, a farmaci ad effetto placebo; Noi oggi siamo davanti ad un malato grave, gravissimo, quasi terminale;

ci si affida ad un ennesimo tentativo, che magari può anche essere considerato un effetto placebo o una pozione magica. Lo dico con molta chiarezza:

La Commissione si è assunta la responsabilità, ad esempio all'articolo 2 (che questo Parlamento ha votato), nella parte che riguardava il delicato rapporto con la magistratura, di scrivere un

dicendo loro di occuparsi innanzitutto della raccolta differenziata e dell'impiantistica, pensando ad esempio alla localizzazione degli impianti di compostaggio.

per fare in modo che sia finalmente approvato un piano regionale per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti. Senza questo piano, noi passeremo di venti giorni in venti giorni, da discarica a discarica, da rivolta a rivolta, da emergenza a emergenza, fino a che questo non sarà più possibile farlo, perché

ma anche quella di poter finalmente varare e consegnare il piano regionale dei rifiuti, altrimenti non c'è davvero alcuna speranza

Sono stato tentato di riproporre, senza cambiare una sola virgola, l'intervento che ho pronunciato in quest'Aula non più tardi di sei mesi fa quando, con analogo atto di Governo,

A questo proposito, va dato atto a Bertolaso che almeno qualcosa ha fatto: ha ridotto gli sprechi dei mega-affitti e ha individuato una sede già dello Stato; ci sono voluti 14 anni per fare questo, però ha cominciato con qualche risparmio. Non si direbbe che sia passato tanto tempo. È ben vero che non si poteva chiedere a Bertolaso di risolvere in nove mesi ciò che altri non hanno risolto in 12 anni,

«Qui non si tratta di voltare pagina, ma si tratta di scrivere un nuovo libro». Noi di questo nuovo libro non abbiamo visto niente: né l'indice né l'inizio. Abbiamo rivisto le stesse scene di cumuli di spazzatura, di cassonetti dati alle fiamme, di proteste della popolazione contro la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e lo stesso sprezzante disinteresse da parte delle istituzioni locali - presidente della Regione Bassolino in testa - che attendono che altri risolvano il loro problema. Nel frattempo, lo Stato getta via 200 milioni di euro l'anno per le soluzioni tampone che possono chiamarsi stoccaggi o viaggi all'estero delle "scoasse", come si dice in veneto. Altro sospetto Altro sospetto è che ci sia da parte di alcuni un disegno preciso che porta cinicamente a sfruttare l'emergenza, e la cronaca delle ultime settimane alimenta questo sospetto: in pochi giorni sono stati allontanati uno dopo l'altro i due subcommissari nominati da Bertolaso su indicazione di referenti politici locali. Il primo, dicono i giornali, è stato anche arrestato dalla Guardia di finanza nell'ambito di un'inchiesta su tangenti e criminalità organizzata nel settore rifiuti. Nel frattempo - ma era inevitabile che accadesse, in un lasso di tempo così lungo - si sono formati all'interno del commissariato dei veri e propri centri di potere che fanno letteralmente il bello e il cattivo tempo: prima decidono quali sono i Comuni da privilegiare per lo scarico dei rifiuti, cioè chi merita di avere le strade pulite e chi no (e casualmente chi ha le strade pulite sono tutti Comuni di centro-sinistra), poi decidono quali fornitori pagare e quali no, assicurando comunque regolari rimesse alla FIBE e alla sua catena di subfornitori, alcuni dei quali notissimi nelle cronache criminali.

siti per gli impianti di smaltimento, cosa fa? Incarica l'azienda municipale di gestione dei rifiuti di bandire una gara esplorativa per lo smaltimento fuori Regione dei rifiuti. Guarda caso, al vertice dell'ASIA siede oggi l'ex vice commissario all'emergenza rifiuti che evidentemente ha in animo di realizzare un commissariato parallelo o - chissà ? - di preparare il terreno per quando, a fine anno, scadrà il mandato Bertolaso. Una cosa deve essere evidente: non è tollerabile che si pensi per il 2008 ad un rinnovo dell'emergenza. I cittadini italiani sono stufi di pagare per l'inefficienza della Campania. Ha ragione Fassino quando dice che i cassonetti in fiamme hanno fatto perdere al centro-sinistra più voti a Como che non in Campania. E a questo proposito ho sentito

Governo, onorevoli colleghi, la posizione del nostro Gruppo è stata espressa in discussione generale in modo chiaro ed articolato dal senatore Bellini, che ha ricordato come non avremmo voluto qui discutere il terzo decreto speciale, in due anni, per la Campania. Dal febbraio 1994, anno della prima dichiarazione dell'emergenza, ad ora sono passati quasi ben 14 anni, e dopo tutto questo tempo non può più esserci nulla di straordinario: c'è una responsabilità della politica in tutto questo. questo. Nella vicenda campana, se una cosa è mancata, è la buona politica; quella fatta di confronto, di partecipazione, di discussione ed anche di contrasto, dove occorre; la politica capace di rappresentare gli interessi della comunità e di portarli a mediazioni ed a sintesi condivise. La politica è stata sostituita dalla legittimazione di una persona ed abbiamo visto come il potere formale, senza la legittimazione sostanziale data dal consenso faticosamente cercato e costruito tra i cittadini, è un vuoto simulacro. Vasti poteri commissariali si sono ridotti a mera apparenza ed hanno prodotto, alla fine, solo ritardi. È così che si pongono le premesse della protesta, del rifiuto da parte delle comunità locali di oneri che, altrimenti, davanti a sacrifici equilibrati e condivisi, bene si potrebbero chiedere che fossero accettati. Alla politica dei cittadini è rimasto solo lo scontro di piazza. Le istituzioni sono rimaste isolate e si sono mostrate sorde ed autoreferenziali. Qui troviamo la responsabilità dei soggetti politici fino al punto che scelte, davvero cruciali, sono state affidate e poi lasciate, addirittura, a soggetti privati. Dove sono in questo modo i fondamenti di un sistema democratico? Quali interessi sono rappresentati e da chi? Chi risponde a che cosa? In quale sede? La vicenda campana è l'esempio della politica che noi non vogliamo: che sia di insegnamento! Noi speriamo che si avvii concretamente, con questo decreto, l'uscita dall'emergenza, il ritorno alla normalità, non solo con una formale definizione dei poteri ma anche e, soprattutto, nella sostanza, con il recupero, proprio e fisiologico, da parte dei soggetti politici, delle istituzioni, delle sedi proprie, della partecipazione popolare. Noi voteremo a favore, ma da quanto ho detto è chiaro che non votiamo per la cattiva politica; non votiamo per gli errori fatti, per le mancanze evidenti, passate e presenti. Il nostro voto esprime la nostra piena solidarietà non ai governanti della Campania ma ai governati, alle donne ed agli uomini della Campania, che devono essere oggi difesi nel loro diritto alla salute e ad un ambiente dotato di salubrità. Noi votiamo a favore perché non accada più in futuro di apprendere che le statistiche sanitarie di una delle maggiori Regioni del nostro Paese sono drammaticamente volte verso il basso. Il nostro voto favorevole è per i cittadini, per gli uomini e le donne della Campania.

al senso di responsabilità, ma quello che mi meraviglia è anche l'ultimo intervento del presidente Salvi quando dice: «Non avremmo voluto votare un altro decreto Campania».

l'articolo 1 va in deroga a tutte le norme di tutela della salute dei cittadini; l'articolo 2 lega le mani alla magistratura che vuole tutelare quei cittadini; l'articolo 4 obbliga economicamente i Comuni ad usare i consorzi, senza sapere quanto verrà a costare, pagando quelle spese create in tutti questi anni; l'articolo 7, caro Salvi, carica sui cittadini della Campania i costi di questa operazione, così come con l'articolo 8 non avete voluto dare una copertura a tutta quella nefandezza che state facendo. Poi c'è

e si fa anche interprete dei tanti, e lo hanno dichiarato anche poco fa, che nella stessa maggioranza sono delusi, che hanno votato solo perché fanno parte di una maggioranza che non sta in piedi se mancano due voti.

Tanti nella maggioranza hanno buon senso ma non lo possono dire, perché quella di cui abbiamo discusso in questi due giorni è solo una questione di buon senso. Qui l'unica cosa che è mancata è proprio il buon senso. Ho girato la Campania e continuerò a girarla insieme al presidente D'Onofrio per spiegare quanto è accaduto in quest'Aula, per spiegare che è stata difesa una classe dirigente che ha fatto solo danni, che non è riuscita in tanti mesi, in particolare negli ultimi 6-7 mesi di gestione commissariale a trovare siti idonei per risolvere i problemi. Una classe politica che - caro senatore Salvi, lei lo chiede da tempo - non si assume la responsabilità di governare. Quella Quella classe politica che avete difeso qui e che continua a spendere i soldi, non difendendo i cittadini, ma aprendo sedi a New York, facendo gite in giro per il mondo o dando consulenze, che sono tantissime anche da parte di questa gestione commissariale. Tutto ciò mentre i cittadini campani devono pagare e tacere; ma allora non dovreste chiamarli cittadini ma sudditi. Continuiamo così. Non ci rallegriamo di quanto è accaduto oggi. Siamo veramente molto tristi, perché ancora una volta avete e abbiamo perso un'occasione. Ha perso questa Aula, che si è adeguata a un Governo che sopravvive e ad un commissariato che a sua volta si è adeguato a questo Governo. Siamo molto più tristi, perché purtroppo, ancora una volta, al di là di quello che viene detto in giro per le piazze campane, hanno perso i cittadini campani, che ancora oggi - forse avete sentito qualche trasmissione in diretta - sono profondamente delusi. È un'altra brutta pagina della politica, ma noi, ricordatevelo, pur considerandola brutta, non siamo rassegnati e continueremo in questa battaglia in modo ancora più energico.

Confalonieri, e anche per la pazienza e il lavoro di miglioramento di questo decreto al quale ha contribuito il sottosegretario D'Andrea. Siamo riusciti, al termine di queste tre settimane di lavoro, a licenziare un testo decisamente migliore di quello che era entrato in quest'Aula. Credo anche che il dibattito abbia contribuito a chiarire gli elementi che hanno portato alla situazione di nuova, ennesima emergenza nella Regione Campania.

ha ricevuto e riceve ancora, in queste ore, tantissimi rifiuti tossici e nocivi che sono frutto delle aziende del Nord, che preferiscono i trafficanti illeciti piuttosto che il ciclo ordinario e legale

un elemento di chiarezza rispetto alle molte inesattezze che ho qui sentito. I laghetti della morte del litorale domizio, che sono stati inquinati fin nelle falde profonde dai bidoni tossici rivenienti rivenienti dai traffici illeciti, sono la tragica dimostrazione del tasso di inquinamento e di mortalità più alto dell'intero Paese, come ci rappresenta l'Organizzazione mondiale della sanità. Questo non è il frutto solo dell'inefficienza, rispetto alla quale chi parla non è stato mai tenero. Il Gruppo che rappresento non è stato mai tenero neanche nei confronti della Giunta regionale di cui il mio partito faceva e fa parte.

della Regione Campania completamente diversa. Allora, credo che sia servito e serva ancora in queste ore compiere un'operazione di verità. Oggi abbiamo davanti a noi un'esigenza, cui credo che il decreto risponda: in primo luogo, dobbiamo liberare le strade della Campania dai rifiuti uscire dall'emergenza, ma abbiamo posto dei paletti ben chiari. Dopo l'attuale emergenza, mai più emergenza e rientro alla gestione ordinaria, perché la gestione commissariale ha alimentato

di pretestuosità e di mistificazione della realtà perché - lo ricordo a me stesso e al senatore Sodano - stiamo parlando della fase delicata (è l'unico riferimento che faccio al passato e che sono costretto a fare) di passaggio tra il Governo Rastrelli e il Governo ribaltonista di Losco, che determinò il rapporto con la FIBE e la possibilità che la FIBE sottoscrivesse il contratto

che queste cose le conosce bene, anche perché oggi sta al Governo con i ribaltonisti di allora, vorrei ricordargli ed evidenziargli che questo decreto è in alcuni punti pericolosamente eversivo, in altri pericolosamente invasivo e in altri ancora pericolosamente evasivo. Si tratta, comunque, di una metafora del grande fallimento delle istituzioni, della politica e del sistema campano: dal rinascimento annunciato al fallimento dichiarato, da «La montagna di sale» di Mimmo Palladino alla montagna di rifiuti di Antonio Bassolino, dall'arte contemporanea al disastro quotidiano, dall'eccellenza all'emergenza; «Miseria e nobiltà» o, se si preferisce scendendo più a Sud, «Così è se vi pare»; Eduardo, Pirandello e Pulcinella, la maschera che si maschera per la vergogna. Si racconta perfino che il Vesuvio abbia un po' di nervosismo e di turbamento perché teme di ritrovarsi, con la montagna di rifiuti, un maleodorante dirimpettaio. Divagazioni? Credo si tratti piuttosto di frammenti di realtà, di immagini per raccontare "a nuttata ca nun passa" e che questo decreto non contribuisce ad illuminare. Abbiamo la lacerante consapevolezza delle difficoltà e della drammaticità della situazione

che ci conferisce il diritto alla chiarezza e alla durezza delle argomentazioni e delle contestazioni e alla nettezza della proposta alternativa per cambiare il senso e l'impostazione di questo provvedimento,

e con la relazione stralcio della Commissione d'inchiesta sui rifiuti, ne avrebbe colto la schizofrenia e la confusione istituzionali, perché tale decreto detta un'impostazione esattamente diversa rispetto a quella della legge regionale. La legge regionale della Campania, sottolineata come evento storico,

di quelle quattro discariche previste al primo punto: in realtà, tutto è stato costruito per approvare un decreto in relazione ai siti addirittura di un decreto *ad situm* - per aggredire Ariano Irpino che, solo attraverso il recupero di un ruolo minimo della politica nel dialogo duro e forte con i soggetti coinvolti, ha determinato un passo indietro rispetto all'arroganza del Governo, respinta dalla mobilitazione delle coscienze e delle istituzioni. Per fortuna, c'è un'altra Campania,

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo Forza Italia voterà contro questo decreto che parte dalla constatazione, ahimè sotto gli occhi di tutti, di un'incredibile emergenza. La affronta, tuttavia, in maniera assolutamente frammentaria e schizofrenica, attraverso interventi

il diritto di individuare i siti, ma, durante la discussione in Parlamento, riconosce di non aver neanche le risorse per poter compensare i Comuni interessati da quell'individuazione e, con la complicità della maggioranza, elimina anche la previsione, per quanto ipotetica fosse, di poter intervenire sulle compensazioni ambientali in quei Comuni dove insistono quei siti. Ciò è assolutamente grave

o forse maliziosamente non voglia quantificare, l'esatto importo degli interventi emergenziali ribaltandone la determinazione e, quindi, l'onere direttamente sui cittadini campani.

Certamente, non vorremmo essere nei panni di un commissario straordinario obbligato a muoversi senza una determinazione esatta di fondi e ad intervenire sulla libera determinazione delle istituzioni locali, mettendo le mani nelle tasche dei cittadini campani per sovvenzionare attività che dovrebbero essere a carico dell'erario.

auspicato che quello fosse l'ultimo decreto di tal genere e che, finalmente, si procedesse ad un ritorno alla normalità e ad una gestione razionale dei rifiuti in Campania, come accade in tante altre aree del nostro Paese.

all'aiuto dei colleghi dell'opposizione (penso ai senatori Libé, Viespoli, Izzo e allo stesso senatore D'Alì), di cui abbiamo accolto molti emendamenti per migliorare questo decreto-legge: credo che siamo riusciti abbiamo occupato molto tempo anche in quest'Aula con discussione di questo decreto-legge. Capisco, quindi, l'esasperazione di molti colleghi, anche della maggioranza, ma non dobbiamo fare l'errore di confondere la causa con l'effetto. Questa successione di decreti è l'effetto di una situazione che si trascina ormai da quattordici anni. Ai colleghi deve essere chiaro che le responsabilità della situazione sono diffuse, sono di un'intera classe dirigente, specialmente campana, che ne porta per intero la responsabilità, ma dovute anche a sottovalutazioni nazionali che hanno accompagnato per quattordici anni questa situazione, questo disastro squisitamente locale. locale. È verissimo, come ricordava il presidente Sodano, che la situazione attuale nasce da una diffusa criminalità organizzata, dalla gestione della camorra

cari colleghi, provenivano da tutti gli schieramenti politici. Il primo fu un commissario di centro-destra ed è lui che porta la responsabilità di quell'accordo con la FIBE gran parte della colpa di cui oggi paghiamo le conseguenze. Ricordiamo la responsabilità della grande impresa

mostrano per intero la responsabilità di un fallimento grave, come quello causato dalla FIBE e da quello che ha fatto in questi anni. anni. Va bene l'autoflagellazione della classe politica, che in questo caso è quanto mai sacrosanta, ma ricordiamoci che le responsabilità sono di un'intera classe dirigente e quindi anche dell'impresa e dell'impresa privata che malissimo si è comportata in Campania nella gestione dei rifiuti. rifiuti. Non voglio però negare (come non hanno fatto molti dei miei colleghi dell'Unione) che le responsabilità siano anche del centro-sinistra, di quei commissari che provenivano dalle nostre file che si sono succeduti in questi anni, a cui è mancato il coraggio di cambiare radicalmente strada, di cambiare lo spirito e le concrete soluzioni - peraltro irrealizzabili - che quel piano stesso conteneva: bisognava cambiarlo, e non è stato fatto.

collocazione e localizzazione di termovalorizzatori, come ricordava il collega Zanone, ma si sono persino battuti contro la collocazione e la realizzazione degli impianti di compostaggio, degli impianti di compostaggio, assolutamente necessari per concludere il ciclo dei rifiuti e realizzare quella frazione

abbiamo vissuto una giornata intensa e non abbiamo ancora ricevuto risposta rispetto alla questione sollevata stamane sulla vicenda Visco. Abbiamo chiesto di sapere se c'è un atto se c'è un atto di revoca delle deleghe, se tale atto è stato o meno pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, se c'è un procedimento corretto o se invece è tutta una finzione che consente a Visco di esercitare poteri che non dovrebbe avere. Signor Presidente, c'è un'altra questione poi sulla quale volevo richiamare la sua attenzione.

si è lamentato di non essere stato avvertito dell'operazione di fusione visto che due Ministri avevano chiesto verifiche sulle indiscrezioni che circolavano sulle operazioni.

e se non si ritenga che tale comportamento rappresenti una grave violazione del principio di'indipendenza e di separatezza che dovrebbe regolare i rapporti tra potere politico e autorità indipendenti rispetto ad operazioni sensibili, con riflessi sui mercati finanziari. Presidente, richiamo infine un'altra questione di più grande attualità. Oggi sono state presentate le tracce dei temi per la maturità. È avvenuto un fatto grave: una scelta giusta come quella della traccia dantesca si è rivelata sbagliata nel modo in cui è stata illustrata. Con superficialità ed approssimazione si è determinato un errore grave che ha portato e porterà molti studenti che hanno scelto quella traccia a sbagliare: con un percorso errato sono stati portati fuori strada, così come tutte le decisioni del Governo di questi giorni. Mi chiedo quale sarà il giudizio del figlio del ministro Fioroni su questa scelta sbagliata.

sull'eventuale esistenza di un decreto di revoca delle deleghe al vice ministro Visco. Ho presentato oggi un'interrogazione. Poiché un giornale riporta una

continuità - non posso che richiamarmi a quanto ha riferito all'Assemblea non molto tempo fa il presidente Marini, dicendo che avrebbe assunto informazioni a fronte delle richieste di specificazione rispetto alle deleghe; quindi, ovviamente, il presidente Marini riferirà nei modi